Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 10 aprile 2015 Onorevole Presidente, informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Vice Ministro al Ministero dello sviluppo economico rassegnate dal prof. Claudio DE VINCENTI e, con ulteriore proprio decreto, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato il medesimo prof. Claudio DE VINCENTI Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo,

recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

il decreto-legge n. 7 del 2015, come modificato a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di 21 articoli, ripartiti in cinque capi. finalizzato al contrasto al terrorismo internazionale, nonché alla proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il provvedimento è stato assegnato all'esame delle Commissioni riunite giustizia, difesa e affari esteri in data 1º aprile, ovvero a pochi giorni utili di attività del Senato rispetto alla data di scadenza per la conversione. Pertanto di fatto, signor Presidente, il contributo ad un atto così importante, che modifica in modo significativo il nostro ordinamento giuridico, è stato relativo, non avendo potuto avviare un proficuo dibattito politico. Si tratta di un decreto-legge che innova il codice penale, con nuove fattispecie di reato per l'emersione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, che modifica il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario, così come il codice antimafia e il codice per la tutela della *privacy*, che modifica ed amplia l'azione dei Servizi di informazione e sicurezza e che istituisce la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Il provvedimento si è reso necessario per introdurre nel nostro sistema misure urgenti di contrasto al terrorismo internazionale, contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, anche in attuazione della risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vincolante per gli Stati, finalizzata all'adozione di misure di prevenzione e di emersione del fenomeno, elevando a reato anche gli atti cosiddetti preparatori e gli spostamenti spostamenti mirati alla partecipazione ad atti di terrorismo. È indubbio infatti che il quadro di legalità e di sicurezza internazionale sia in continua evoluzione nell'area di crisi del Mediterraneo allargato dal 2011 ad oggi e che la minaccia alla sicurezza sia estesa all'Europa. Ce lo testimoniano i gravi fatti di Parigi, l'attacco armato alla redazione di «Charlie Hebdo» e al supermercato Hyper Cacher, intorno alle cui vittime si è stretta l'intera coscienza europea, pubblica e privata, trattandosi di un attentato alle libertà fondamentali della nostra democrazia. L'attacco al museo di Tunisi, che ha coinvolto anche nostri cittadini, ha reso ancor più evidente una minaccia senza confini e che segue schemi nuovi di formazioni terroristiche e di interventi che si avvalgono di gruppi locali, di singoli combattenti

il rispetto dei diritti dell'uomo, la lotta al finanziamento del terrorismo, legato anche al riciclaggio di denaro, una rafforzata capacità di crescita economica e sociale in quelle aree, il consolidamento dei processi di democrazia rappresentano pertanto facce di un unico aspetto, complementari e che si rafforzano vicendevolmente. Il terrorismo islamista va dal *jihad* afgano all'Islam radicale, dall'11 settembre 2001 ad oggi, tra nuove organizzazioni e nuovi sodalizi, da Al Qaeda e al-Zarqawi fino alla alla proclamazione, da parte di Abu Bakr al-Baghdadi, della rinascita del califfato e di uno Stato islamico fondato su violenza e crimini internazionali contro l'umanità, persecuzioni di minoranze e milizie che procedono con lapidazioni, decapitazioni, uccisioni efferate, trafficanti di morte e di esseri umani, da Boko Haram in Nigeria e Kenya, fino alle fosse comuni di Tikrit e ai campi profughi di Yarmouk; violenza indiscriminata nelle scuole come negli ospedali, sino alla distruzione di opere architettoniche e artistiche e di un patrimonio archeologico simbolo di civiltà e cultura. In tale grave contesto si è reso necessario perciò rafforzare gli strumenti interni di contrasto al terrorismo, innovando il nostro ordinamento giuridico con il decreto-legge n. 7 del 2015. Il capo I (articoli da 1 a 8) detta disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale. In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i cosiddetti *foreign fighters*, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e si applica salvo che non ricorrano la più gravi fattispecie della partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo. Inoltre, prevede una nuova fattispecie per chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo, mentre l'articolo 270-*quinquies* punisce colui che, dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi, cosiddetto autoaddestramento, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti. La pena è aggravata per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Inoltre, è previsto che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegua l'obbligo della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale «quando è coinvolto un minore». L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei cosiddetti *foreign fighters*. Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Analoghe aggravanti sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, delitti per i quali viene previsto ora l'arresto obbligatorio. In materia di intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, si prevede la possibilità di utilizzare programmi informatici per acquisire da remoto le comunicazioni e i dati presenti in un sistema informatico. Viene modificata, poi, la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale: per autorizzare le cosiddette intercettazioni preventive anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche; per stabilire che il procuratore della Repubblica che ha autorizzato le intercettazioni preventive, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione consente la conservazione dei dati di traffico acquisiti per un periodo massimo di ventiquattro mesi; tale deroga non include, naturalmente, i contenuti delle intercettazioni; per ammettere, in ogni caso, l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, con il consenso tuttavia del legittimo titolare. La polizia postale e delle comunicazioni dovrà altresì costantemente tenere aggiornata una *black list* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura. Previa richiesta dell'autorità giudiziaria e preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, sono introdotti in capo agli Internet *provider* specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete, di cui dovrà rendere conto il Ministro dell'interno in un'apposita sezione della relazione annuale sull'attività delle forze di polizia. Inoltre, si dispone che il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni in materia di armi: la detenzione abusiva di precursori di esplosivi, sensi del regolamento UE 98/2013, nonché la mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori per le condotte previste dal regolamento di cui sopra. Una sanzione amministrativa è prevista invece a carico degli operatori che, legittimamente trattando tali sostanze, omettono di segnalare operazioni sospette alle autorità, e vengono imposti obblighi di comunicazione a chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplodenti, per consentire al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia, per il tramite delle questure per via informatica o telematica. Il testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) viene inoltre modificato per prevedere: obblighi di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata capienza di colpi; la detenzione abusiva di armi, la violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori è quindi punito a titolo di contravvenzione. La denuncia dei citati caricatori di armi dovrà essere effettuata entro il 4 novembre 2015. Inoltre, viene introdotto un divieto un divieto nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria di cui alla direttiva UE 91/477 e viene dettata una disciplina transitoria relativa all'uso delle armi escluse dall'uso venatorio. L'articolo 3-*bis* integra, inoltre, l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e l'articolo 380 del codice di procedura penale. Con la prima modifica si prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia (ed è previsto l'arresto obbligatorio). L'articolo 4 interviene sul codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per estendere la disciplina delle misure di prevenzione e di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo, applicate dall'autorità giudiziaria, e viene introdotto un provvedimento d'urgenza del questore che, già in sede di proposta al tribunale della misura di sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, possa disporre nei confronti del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento di identità. Viene altresì estesa al procuratore nazionale antimafia, ora anche antiterrorismo, la titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. La commissione di delitti in materia di terrorismo nel corso dell'applicazione di misure definitive di prevenzione comporta l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena, ed è previsto un nuovo delitto relativo alla violazione del divieto di espatrio. Nel testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) è introdotta l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche. Infine, nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale viene raddoppiato, da cinque a dieci giorni, il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cosiddette preventive presso il pubblico ministero che le ha autorizzate. L'articolo 4-*bis* modifica l'articolo 132 del codice della *privacy* in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telematico

L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, nonché la legge sull'ordinamento penitenziario, al fine di estendere la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia e di indagini Si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i Servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi, su richiesta del Presidente del Consiglio e su autorizzazione del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, di cui deve essere informato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e ne è data informazione anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Viene richiamata l'applicabilità della disciplina derogatoria dell'obbligo di denuncia dei reati nonché la possibilità, per i direttori dei Servizi di informazione di ritardare la comunicazione all'autorità giudiziaria degli elementi di prova acquisiti in ordine alla commissione dei reati. Anche in tali ipotesi, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. L'integrazione del contenuto dell'art 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di colloqui prevede la possibilità per il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di svolgere, senza autorizzazione, colloqui investigativi con i detenuti; al medesimo procuratore vanno comunicati i provvedimenti di autorizzazione ai colloqui con persone indagate, imputate o condannate per delitti con finalità di terrorismo. L'articolo 6*-bis* modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia per coordinarne il contenuto con il ruolo del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, cui spetterà, ai sensi dell'articolo 11, la proposta di ammissione alle speciali misure di protezione per la revoca o sostituzione della custodia per l'applicazione di benefici penitenziari. L'articolo 6*-ter*, inoltre, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007, contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per prevedere che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. L'articolo 7 interviene sul codice della *privacy* n. 196 del 2003) per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia, non solo quando il trattamento per finalità di polizia sia previsto dalla legge, ma anche quando sia previsto da una norma regolamentare. L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna. È anzitutto modificato l'articolo 497 del codice di procedura penale per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte sotto copertura, possa fornire le generalità di copertura usate nel corso delle operazioni autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. Inoltre, si attribuisce anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione. è affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Delle citate attività, il Presidente del Consiglio dei ministri informa mensilmente il Copasir. Gli articoli 9 e 10, infine, che compongono il capo II, relativo al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedono l'attribuzione al procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti organizzativi, in tema sia di contrasti tra pubblici ministeri, che di trasmissione degli atti ad altro pubblico ministero per incompetenza, prevedendo l'accesso del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo al registro delle notizie di reato, ai registri delle misure di prevenzione e alle banche dati istituite appositamente presso le procure distrettuali, nonché alle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti con modifica alcuni articoli del codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo istituita nell'ambito della procura generale della Corte di cassazione. Signor Presidente, prima di passare la parola ai colleghi senatori relatori sul capo III,

proposta dalla 14a Commissione sulle politiche europee nel Mediterraneo. Infatti, davanti alla grave instabilità che coinvolge una vasta area del Mediterraneo e del Medio Oriente, occorre insistere affinché sia l'Unione europea nella sua unità ad elaborare risposte comuni (oltre che a modificare gli ordinamenti interni), interni), politicamente forti ed efficaci, per una nuova ed aggiornata strategia di sicurezza europea; occorre, altresì, restituire centralità e priorità alla frontiera unica europea sul Mediterraneo, in termini di sicurezza, ma anche di opportunità, di solidarietà e di controllo. Insomma, occorre un nuovo paradigma per un quadrante strategico, del Mediterraneo allargato, la cui stabilità politica, la cui crescita democratica, economica e sociale ci riguardano, come protagonisti. Oggi ancor di più un'assunzione di responsabilità è dovuta.

per quanto di competenza della Commissione esteri, il disegno di legge in esame, proroga, fino al 30 settembre 2015, le missioni internazionali in corso e gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione. Il provvedimento conferma l'approccio multilateralista tradizionale del nostro Paese, che sostiene quelle attività e missioni attraverso cui la comunità internazionale punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia si connota peraltro per uno sforzo volto a coniugare la dimensione militare con quella civile, per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una duratura stabilizzazione nelle principali aree di intervento. con il presente decreto viene confermato, affiancando alle missioni in senso stretto interventi ed iniziative in ambito umanitario, di rafforzamento dello stato di diritto, di sostegno alle amministrazioni locali e alle strutture di governo e di miglioramento economico e sociale. Il capo III del provvedimento conferma l'autorizzazione di spesa, sino al 30 settembre 2015, per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, che sono suddivise sulla base di criteri geografici, a partire da quelle in Europa, di cui all'articolo 11 (Georgia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Cipro e Mediterraneo), Asia, di cui all'articolo 12

Di rilievo anche la disposizione contenuta nell'articolo 14 che autorizza per l'anno 2015 una spesa complessiva di circa due milioni di euro per interventi urgenti di prima necessità delle popolazioni locali nei casi di necessità ed urgenza disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipino alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa e Libia. Tra le altre previsioni di interesse nel capo III si può segnalare la decisione di subordinare il prosieguo della operazione militare dell'Unione europea antipirateria denominata Atalanta una volta conclusa e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015 - alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina, sentite in ogni caso le competenti Commissioni parlamentari (articolo 13, I profili di specifico interesse per la Commissione esteri sono contenuti nel capo IV del testo, relativi ad iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17), al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18), al regime degli interventi e altre disposizioni per l'operatività dell'amministrazione del Ministero degli esteri (articolo 19) e alla materia della sicurezza dei viaggiatori (articolo 19-*bis*). L'articolo 17 autorizza sino al 30 settembre una spesa di 68 milioni di euro - ad integrazione degli stanziamenti già previsti nella legge di stabilità 2015 per iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in una serie di Paesi: Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, oltre che per l'assistenza ai rifugiati nei Paesi limitrofi. È previsto altresì che il Ministro degli esteri e della cooperazione agevoli l'intervento di organizzazioni non governative nei Paesi richiamati, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività (comma l-*bis*, articolo 17). Tali interventi, che il Ministero è tenuto a rendere pubblici, devono avere particolare attenzione su alcuni temi: la tutela dei diritti delle donne (ed in particolare contro la violenza di genere), dei minori, degli anziani lo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute e il contrasto all'epidemia del virus Ebola. È poi prevista una spesa di 1,7 milioni euro per attività di sminamento umanitario (articolo 17, L'articolo 18 autorizza per il 2015 l'erogazione di un contributo di 120 milioni di euro a supporto delle forze di sicurezza dell'Afghanistan, incluse le forze di polizia. Il medesimo articolo (al comma 2) destina una somma complessiva di quasi 1,5 milioni di euro ad interventi a sostegno della stabilizzazione in Paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto: principalmente Libia, Siria e Iraq. Ulteriori due milioni di euro sono poi destinati alla realizzazione di interventi ed iniziative a sostegno dei processi di pace nei Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America latina e caraibica. Sono inoltre previsti 2,3 milioni di euro per la partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale per il Libano e alla costituzione di un fondo per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (con una dotazione di 500.000 euro). Gli ulteriori commi dell'articolo autorizzano: una spesa di circa 10,8 milioni di euro per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario dell'INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e alla Fondazione segretariato permanente dell'iniziativa adriatico-ionica (al comma una spesa di circa 9,2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero una spesa di 23 milioni di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti italiani di cultura e scolastici all'estero, nonché per assicurare condizioni di sicurezza per il personale impiegato in aree di crisi Lo stesso articolo 18 autorizza poi una spesa di 700.000 euro per gli interventi di realizzazione della nuova sede dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio (comma 8),

L'articolo 19 contiene poi una norma di salvaguardia degli atti e delle attività già svolte dal 1 gennaio 2015 che risultino conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge in esame e nei limiti delle risorse stanziate. L'articolo prevede altresì (al comma 2-*bis*) che il Ministero degli esteri possa collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, sospendendo in tal caso la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti. Da ultimo l'articolo 19-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce al Ministero degli esteri e della cooperazione la funzione - che in realtà già svolge - di rendere pubblici, tramite il proprio sito, le condizioni e gli eventuali rischi per i viaggi in Paesi stranieri, indicando altresì comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.

il decreto-legge posto in votazione risente della ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento dovuti alla imminente scadenza. Ringrazio quindi da subito gli uffici e tutti i colleghi delle tre Commissioni che ha concesso di approdare al dibattito in Aula in tempi brevi. Vi è un contesto straordinario in cui si colloca oggi il nostro compito di legislatori.

indica, quale fondamento normativo dell'intero provvedimento, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e che tratta delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo. La relatrice, senatrice Ginetti, ha delineato e contestualizzato bene il dibattito odierno e l'esame delle singole disposizioni di cui si compone il decreto-legge nella prospettiva del carattere globale della lotta contro il terrorismo. Successivamente, il relatore Maran ha inquadrato altrettanto bene l'approccio multilaterale alla politica estera del nostro Paese. In premessa, quindi, è indispensabile accennare ai profondi sconvolgimenti che si sono succeduti in questo ultimo periodo nello scenario internazionale, all'evidente moltiplicarsi delle minacce alla pace e alla stabilità e al peggioramento delle condizioni di sicurezza che tutti possono riscontrare. La situazione è in continua evoluzione, sta ridisegnando l'intero quadro delle relazioni internazionali e ha un effetto per quanto riguarda la nostra proiezione internazionale. Tuttavia, com'è stato ricordato, è evidente che l'Italia nella sua politica estera e di difesa deve darsi priorità specifiche e bene orientate, tenendo conto della nostra particolare esposizione nei confronti delle crisi presenti nell'area del Mediterraneo allargato. Questo tipo di approccio deve essere confermato anche per il futuro, naturalmente, portando anche la specificità della nostra prospettiva, come ha come ha fatto e continua a fare il Governo, e anche questa Assemblea con il proprio contributo, portando al centro dell'attenzione della politica europea il tema specifico del Mediterraneo. Per quanto riguarda le missioni internazionali, siamo di fronte a una pratica divenuta costante dal 2001, e che riguarda le missioni previste dallo stesso provvedimento entro i limiti temporali da esso stabiliti. È necessario, in questa precisa contingenza, operare scelte calate nel reale contesto delle missioni internazionali in relazione alle svariate implicazioni che da esse discendono. Di più, in mancanza di una disciplina quadro della materia, il ricorso a questo provvedimento risponde alla necessità di adeguare la disciplina normativa alle peculiari esigenze operative connesse con le missioni, assicurando in tal modo una disciplina uniforme da applicare in tutti i casi di partecipazione del personale militare alle missioni internazionali di pace. A questo proposito giova ricordare che alla Camera è in corso l'esame di una legge quadro sulle missioni internazionali da cui possa scaturire un approccio proficuo alla disciplina di questa materia, nella consapevolezza che il quadro delle missioni è mutato radicalmente e progressivamente negli ultimi anni, con ripercussioni che hanno già, e che avranno ancora inevitabilmente di più, effetto sulla politica della difesa e sulla politica estera. L'attenzione in questa sede deve essere incentrata su aspetti precisi e concreti che rappresentano la vera essenza di questo provvedimento, e cioè il fatto che le missioni internazionali hanno come obiettivo la costruzione della pace e vedono le Forze armate impegnate ed esposte a ogni tipo di rischio proprio per contribuire al mantenimento della pace stessa. Tutte le missioni internazionali dell'Italia hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dalle autorità sia politiche che militari dei Paesi in cui hanno operato; inoltre i nostri militari hanno saputo sempre entrare in sintonia con le popolazioni stanziate nei vari teatri in cui si sono trovati a intervenire. Senza contare che quasi tutte le situazioni che hanno reso e che rendono necessario l'intervento militare comportano impegni a lungo termine, che non possono risolversi in un arco temporale caratterizzato da brevità. L'argomento delle missioni internazionali è, dunque, come già detto a più riprese, tra i più delicati, chiamando in causa temi sensibili come la libertà e la vita umana, che richiedono - è da ribadire con vigore - un altissimo senso di responsabilità nell'approccio alla loro trattazione. Senza dimenticare il tributo offerto, anche e soprattutto in termini di vite umane, dai nostri soldati, che è stato altissimo e che ha testimoniato, anche sotto questo aspetto, il valore di eccellenza che da sempre contraddistingue la nostra presenza nel contesto delle missioni internazionali. La nostra partecipazione alle operazioni internazionali non può non richiamare ancora la questione dei due fucilieri di Marina, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, sostenendo la costante azione del Governo, al fine di concludere in termini definitivi una vicenda veramente paradossale. Le Forze armate sono diventate strumenti funzionali alla sicurezza e alla stabilità della comunità internazionale e ciò comporta, dunque e inevitabilmente, il coraggio politico di impiegare lo strumento militare con queste finalità. La sicurezza, quindi, va considerata nella sua interezza e deve poter contare su decisioni politiche rapide e, appunto, coraggiose. In tale quadro sono stati compiuti notevoli cambiamenti di orientamento e di approccio

imminente del libro bianco della difesa, indispensabile per sviluppare gli elementi culturali ed organizzativi che consentano alla Difesa di contribuire in modo organico allo sforzo del Paese per definire la cornice di sicurezza futura. Passando all'analisi del provvedimento, al capo I, che detta disposizioni di contrasto al terrorismo internazionale, vi sono due norme di specifico interesse per la Difesa. L'articolo 5, nel testo risultante dalle modifiche operate in prima lettura, proroga al 30 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego operativo di cui al decreto-legge n. 92 del 2008 sull'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle forze di polizia, incrementandolo di 1.800 uomini per la prevenzione del terrorismo e prorogando anche, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità nelle province della Regione Campania. Un ulteriore contingente militare, pari a 600 unità, garantirà inoltre i servizi di sicurezza del sito dell'Expo 2015. Importanti le modifiche di interesse della Difesa apportate nel corso della prima lettura In particolare, il contingente operante in Campania potrà essere incrementato, a decorrere dal 30 giugno 2015, fino a 300 uomini e l'Arma dei carabinieri potrà anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri

euro, per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, la cosiddetta operazione Mare sicuro, come anticipato dal Ministro della difesa alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento nella seduta del 19 marzo scorso. A fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia risulta, infatti, necessario adottare misure per assicurare la tutela degli interessi nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l'avanzata della minaccia terroristica. L'infittimento delle attività di pattugliamento, condotte nell'area del Mediterraneo interessata dalle principali rotte di comunicazione, determinerà una maggiore protezione in mare, segnatamente in riferimento al rischio di aumento dei traffici illeciti condotti in mare, principalmente il traffico di armi, di possibili infiltrazioni di terroristi nel territorio nazionale, di possibili azioni di matrice terroristica a danno di installazioni *off-shore* e natanti, civili e militari. Tale rafforzamento contribuirà, altresì, alla raccolta di informazioni sulle attività dei gruppi terroristici che, per gli ulteriori sviluppi, vedranno interessati gli organi competenti. Le risorse stanziate consentiranno di incrementare adeguatamente gli assetti dell'ordinario dispositivo aeronavale di sorveglianza per la sicurezza marittima con l'impiego di ulteriori unità navali, con componente elicotteristica, e aeromobili, anche a pilotaggio remoto, e gli eventuali ulteriori assetti di sorveglianza elettronica. Sono poi disciplinate le modalità di utilizzo di droni da parte delle forze di polizia, che comprendono perciò Carabinieri e Guardia di finanza, con finalità di pubblica sicurezza e di contrasto al terrorismo. L'articolo 8, anch'esso modificato dalla Camera dei deputati, introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna. In particolare, una modifica operata dalla Camera attribuisce all'Agenzia di informazioni e sicurezza esterna (AISE) il compito di svolgere attività di informazione, anche tramite ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi anche di natura militare del Paese. Di specifico interesse per la Difesa è il capo III del decreto-legge, composto dagli articoli da 11 a 16, che reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate sulla base di criteri geografici. È confermata la suddivisione delle missioni in tre articoli sulla base della dislocazione continentale dei contingenti (Europa, Asia, Africa), già adottata a decorrere dal 2014. Sono confermati i teatri operativi contemplati dal precedente provvedimento di proroga e sono inserite, come preannunciato nelle comunicazioni date al Parlamento, la Resolute support mission in Afghanistan, missione della NATO che subentra alla missione ISAF chiusa al 31 dicembre ultimo scorso, di natura *no combat*, finalizzata allo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane,

I militari italiani opereranno, nel corso del primo semestre 2015, a Herat, nella regione Ovest. A decorrere dal secondo semestre 2015, come previsto dalla pianificazione NATO, si procederà ad una riconfigurazione riduttiva delle forze presenti nella zona, in vista del progressivo concentramento nell'area di Kabul. Si segnala che, riguardo alla missione, risultano realizzate le condizioni previste dal decreto-legge

di concerto con le organizzazioni internazionali, e alla comunicazione alla Camera. Ebbene, la risoluzione n. 2189 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, atto del sostegno delle Nazioni Unite alla missione. Il Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan hanno sottoscritto a Kabul il 30 settembre 2014 agreement, nel quale sono definiti i termini e le condizioni in cui le forze della NATO saranno schierate in Afghanistan nell'ambito della missione. Tale accordo è stato ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre

È prevista, al riguardo, un'ulteriore autorizzazione di spesa di circa 2,9 milioni per la corresponsione, ora per allora, al personale che ha partecipato alle medesime attività in Iraq e Kuwait, nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014,

La missione, iniziata su richiesta congiunta della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia, motivata dall'insufficiente possesso di capacità e strutture per la difesa aerea autonoma, ha il compito di sorvegliare e identificare tutte le violazioni all'integrità dello spazio aereo della tre Repubbliche baltiche. Alla missione partecipano 14 Stati membri della NATO, a rotazione. Il concorso nazionale inizialmente era stato accordato fino all'aprile 2015; tuttavia, in occasione della recente ministeriale NATO-Difesa, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2015, è stata espressa in quel consesso, su auspicio del Ministro della difesa lituano, e con l'approvazione e l'apprezzamento dell'Assemblea NATO, la disponibilità dell'Italia a prolungare di altri quattro mesi il proprio concorso aereo, portandolo fino al 31 agosto 2015. È da precisare che tale ulteriore permanenza, finanziata peraltro solo in parte dal presente decreto, vedrà la restante parte della spesa ristorata dallo Stato primo richiedente, cioè dalla Lituania. È stata decisa, per le missioni antipirateria, la partecipazione alla sola missione dell'Unione europea Atalanta, con conseguente riduzione del personale impiegato, da 607 a 525 unità, e, per le missioni in Libia, la riduzione del personale impiegato, da 100 a 30 unità. È stata inserita la previsione che condiziona la prosecuzione della missione dell'Unione europea antipirateria Atalanta oltre il 30 settembre 2015 alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di Marina attualmente trattenuti in India, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto per circa 73 milioni il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE. L'articolo reca inoltre una serie di disposizioni per la cessione a titolo gratuito ad altri Paesi di mezzi e materiale militare. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati prevedono un'ulteriore autorizzazione di spesa di due milioni di euro per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed enti militari. L'articolo 15 contiene norme concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica. Sono abrogate, a decorrere dal 1° giugno 2015, le disposizioni relative all'impiego dei nuclei della Marina militare per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana a rischio di pirateria e, conseguentemente, adeguate quelle riferite all'utilizzo di servizi di vigilanza privata per la medesima finalità.

dell'impegno in ambito internazionale comporterà complessivamente una riduzione di spesa a carico del bilancio della Difesa di circa nove milioni di euro. senatori, termino davvero sottolineando che siamo in una fase storica in cui le diffuse instabilità che vediamo nello scenario internazionale hanno ancora più bisogno di risposte concertate e multilaterali il nostro Paese intende assicurare la sua partecipazione alle iniziative comuni nei confronti delle crisi di oggi. L'Italia è impegnata generosamente in operazioni legate al ristabilimento della pace, della sicurezza e dello sviluppo dei popoli oppressi. In un contesto internazionale segnato dal rompersi di vecchi equilibri geopolitici si riaffermano ancora i principi cardine della nostra politica estera e di sicurezza, la partecipazione ai processi di pace e la conferma del ruolo internazionale del Paese anche nel quadro di grandi operazioni multilaterali.

presentare una questione pregiudiziale perché riteniamo che questo provvedimento abbia molteplici profili di incompatibilità con varie norme costituzionali. Per certi versi anche la stessa tempistica

pare che nell'ordine di pochissimi giorni o forse anche nello stesso giorno, siano stati arruolate più di 2.000 persone per dare un supporto proprio all'attività antiterroristica. Riteniamo vi siano ulteriori perplessità sul fatto che lo stesso provvedimento tratti due materie che avrebbero benissimo potuto essere trattate con due provvedimenti a parte, uno sulle misure antiterroristiche ed un altro sulla proroga delle missioni militari. Cogliamo l'occasione anche per sottolineare che, per l'ennesima volta in un decreto-legge, si vanno ad inserire modifiche che riguardano il codice penale ed il codice di procedura penale. La decretazione d'urgenza non è lo strumento più adatto per

Signor Presidente, anche noi, come già alla Camera dei deputati, abbiamo presentato una questione pregiudiziale perché riteniamo che questo provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, presenti una serie di profili d'incompatibilità, non soltanto con molte norme costituzionali, ma anche con la giurisprudenza costituzionale, che più volte è intervenuta in merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno lo strumento del decreto-legge. Questo decreto-legge, in particolare, presenta una serie di contenuti a nostro avviso assolutamente non omogenei, in quanto accosta la materia del contrasto al terrorismo, anche quello internazionale, a quella delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finanche alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, senza tener conto di diverse indicazioni arrivate nel corso degli anni passati. Mi alla lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica, nella quale si fa riferimento al fatto che provvedimenti eterogenei nei contenuti sfuggono alla comprensione dell'opinione pubblica e rendono ovviamente più complesso il rapporto tra il cittadino e la legge. Va inoltre ricordato il tema secondo il quale i decreti-legge debbano contenere misure d'immediata applicazione ed il loro contenuto debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. possono anche richiamare diverse sentenze della Corte costituzionale, che ha più volte rilevato come i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardino il decreto-legge nella sua interezza, inteso per l'appunto come insieme di disposizioni omogenee

oggettivamente unitario; deve cioè contenere un insieme di disposizioni omogenee, almeno per materia e scopo. Dal nostro punto di vista, basta semplicemente scorrere

che caratterizza il decreto-legge, si è scelto di lavorare su un tema peraltro molto delicato, quale la lotta al terrorismo, con l'introduzione di una serie di nuove fattispecie, appunto con uno strumento, quello del decreto-legge, che evidentemente esplica i propri effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, quindi fin da subito, senza che vi sia stato ancora il vaglio delle Camere. Ora, si capisce bene che, anche dal punto di vista politico,

perché evidentemente ci troviamo di fronte ad un terrorismo particolarmente indiscriminato e crudele, avremmo avuto bisogno di affrontare seriamente il concetto di sicurezza, senza sganciarlo però - come pure rischiamo di fare - dal tema dei diritti e delle garanzie di libertà. Attenzione, perché questo è un tema serissimo; è un tema che ha attraversato la storia della Repubblica italiana nel corso degli ultimi quarant'anni ed è un tema che ha attraversato e attraversa il dibattito politico anche in altri Paesi del mondo, che sono per l'appunto minacciati da elementi terroristi. Evidentemente, il rapporto tra il contrasto al terrorismo

e di grandissima attenzione ed avrebbe meritato, dal nostro punto di vista, un *iter* differente rispetto a quello che è stato scelto, specialmente quando nel decreto in questione vengono allargati i filoni delle fattispecie di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale, ma la materia viene definita, a nostro avviso, in maniera molto poco precisa, peraltro immaginando delle maglie molto larghe, che rendono poco chiara l'individuazione delle problematiche effettivamente presenti. Per di più, il decreto-legge prevede anche un ampliamento dei casi per disporre l'immediata espulsione da parte del prefetto

perché, se trattata in maniera superficiale e se trattata semplicemente in maniera emotiva, emozionale ed emergenziale, può diventare illegittima e finanche criminogena,

antiterrorismo, è previsto anche un ulteriore punto delicato: l'autorizzazione a procedere a colloqui con detenuti ed internati per informazioni circa la prevenzione di reati con finalità terroristica, senza la presenza di un avvocato difensore. Si tratta che a noi sembra molto serio. A ciò si aggiunge l'altra parte di questo provvedimento, che riguarda le missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese. Abbiamo detto più volte nei mesi passati, quando abbiamo affrontato il tema delle missioni, che sarebbe stato molto più serio e più opportuno affrontarle separatamente, perché non è vero che tutte le missioni sono uguali. Ci sono evidentemente missioni che determinano un giudizio politico e un bilancio storico positivo e missioni che invece determinano ben altro giudizio politico; quindi, non fosse altro che per questo, sarebbe stato opportuno discuterle una per una e non tutte quante insieme. Ebbene, in questo caso si continua a discutere delle missioni non in maniera separata.

di riferimento non può però comportare l'obbligo automatico di partecipare ad ogni missione, indipendentemente dal livello di giudizio che il Parlamento nazionale può esprimere nei confronti di ciascuna di esse. Quindi sarebbe stato molto più corretto secondo noi - come non ci stanchiamo di ripetere da molti mesi a questa parte - valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire; invece l'utilizzo dello strumento del decreto-legge impedisce proprio questo tipo di analisi Peraltro, anche le relazioni tecniche che vengono puntualmente allegate ai provvedimenti mancano molto spesso, anche in maniera molto significativa, di tutte le informazioni relative ai costi delle singole missioni. molto azzardato, nella materia data, il richiamo ai requisiti di necessità ed urgenza. Manca, a nostro avviso, anche la caratteristica della straordinarietà dell'intervento governativo, come disposto all'articolo 77 della Costituzione, e per questo proponiamo di non procedere

Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia ha sempre ritenuto estremamente importante la partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali, intendendola

sono importanti perché non possiamo pensare che la prevenzione del terrorismo o degli atti di violenza o di qualsiasi tipo di atto aggressivo nei confronti del nostro Paese possa essere come se fossimo nel XIX secolo, cioè solo schierando gli eserciti ai confini: ovviamente, bisogna avere la lungimiranza e la capacità di sapere che occorre tutelare la pace e determinate situazioni in missioni all'estero. proprio per questo riteniamo estremamente negativo il fatto che il Governo abbia voluto mescolare con questo specifico punto, e cioè quello delle missioni,

opportuna una valutazione approfondita sulle garanzie costituzionali che devono comunque permanere, anche in situazioni di emergenza o di pre-emergenza;

al rischio di una sentenza della Corte costituzionale che un giorno ci dica che quelle misure non sono valide e devono decadere perché sono state varate all'interno di un provvedimento ampiamente disomogeneo. finestra"). Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Diego Valeri» di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il decreto-legge al nostro esame è destinato ad avviare un'adeguata politica di prevenzione e di tutela contro le minacce terroristiche, prevenzione - qui sta il punto - che deve essere effettuata non solo sul piano interno, ma anche su quello internazionale, con particolare riferimento ai territori con maggiore criticità. Nasce da questo l'esigenza anche di norme apparentemente eterogenee, che tuttavia hanno in questo elemento il punto di sintesi e di raccordo. Il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi, infatti, acquisisce sempre di più anche una funzione di carattere preventivo e diviene un elemento essenziale di politica estera con positivi riflessi anche sulla sicurezza dei cittadini. Il contrasto al terrorismo necessita, infatti, di un approccio concreto, responsabile e globale alle questioni che esso pone attraverso misure tese a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione del fenomeno all'interno del Paese e mediante la partecipazione a missioni internazionali che rispondano alle medesima finalità. Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea contiene proprio disposizioni necessarie ed urgenti, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, al fine di contrastare la crescita di un terrorismo che, specie negli ultimi tempi, ha mostrato con una incredibile recrudescenza il suo volto più feroce ed allarmante. In questo contesto diventa, dunque, indifferibile completare il quadro normativo vigente, introducendo misure adeguate e selettive capaci di pervenire il rafforzamento delle organizzazioni terroristiche e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati, per il compimento di attentati, anche nel territorio nazionale. Le disposizioni contenute nel decreto-legge sono, pertanto, rivolte a dare completa attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e, quindi, vincolante per gli Stati. La risoluzione ONU obbliga gli Stati a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso il coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici anche in territorio estero, tema quest'ultimo che riguarda il nostro Paese e le nefaste attività dei *foreign fighter*. Il decreto-legge, peraltro, è collocato proprio all'interno di un contesto che prevede la piena partecipazione dell'Italia all'impegno richiesto dalle Nazioni Unite. È paradossale, colleghi, che venga invocata la pregiudiziale di costituzionalità quando la nostra Costituzione obbliga il nostro Paese, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 11 ad ottemperare alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza proprio in quanto l'Italia, ai sensi di detto articolo, devolve una parte della propria sovranità ad organismi internazionali deputati a garantire un ordine di pace e di giustizia tra le Nazioni. Le norme del provvedimento si ispirano ad una filosofia legislativa unitaria, rappresentata dalla tutela della sicurezza dei nostri cittadini attraverso misure di carattere nazionale ed internazionale. Il Governo quindi, attraverso questo provvedimento, intende porre in essere un'efficace e corretta politica di prevenzione e di tutela contro la minaccia terroristica ispirandosi al principio per il quale questa battaglia, per avere successo, deve essere condotta sul piano della sicurezza sia interna che esterna. Dunque, i profili denunciati dai colleghi di presunta incostituzionalità non hanno ragione di essere. Concludo con un riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013, che riferisce il requisito dell'omogeneità delle disposizioni di un decreto-legge o alla materia o allo scopo. E nella circostanza attuale il profilo dello scopo, cioè la lotta efficace al terrorismo nella sua dimensione interna ed internazionale, è preminente e di difficile contestazione alla luce degli elementi riferiti. È per questa ragione che noi voteremo questo decreto-legge serena coscienza di fare l'interesse del Paese nell'alveo preciso delle disposizioni costituzionali.

Signor Presidente, il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015, che proroga le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e qualche iniziativa di cooperazione allo allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione, viene riproposto senza avere quei requisiti di urgenza che dovrebbero essere propri di questo tipo di provvedimento. Intanto, secondo quanto riportato dalla stampa, la spesa militare italiana è aumentata ancora, passando dai 65 milioni di euro al giorno del 2013 a quasi 70 nel 2014, e tutto lascia supporre che nel 2015 dovrebbe raggiungere gli 80 milioni di euro al giorno. E questo non comprende le spese militari *extra budget*, come quelle che gravitano sul Ministero dello sviluppo economico per la costruzione di sistemi d'arma e sul Ministero dell'economia e delle finanze per il sostentamento delle missioni all'estero. Secondo quanto calcolato dal SIPRI, l'Italia è il dodicesimo Paese al mondo per la dimensione della spesa militare e uno dei più importanti per numero di militari impegnati in operazioni all'estero. Tra le missioni previste dal presente decreto-legge ce ne sono diverse - come, ad esempio, quelle nell'area balcanica - che sono iniziate diversi anni fa, e l'obiettivo iniziale è di fatto mutato: non vi è più la necessità di far rispettare accordi sul cessate il fuoco, ma si effettuano compiti, dal controllo dei confini all'ordine pubblico interno, che potrebbero essere tranquillamente È evidente che quegli Stati hanno interesse a che questi ruoli vengano svolti dalle forze internazionali, consentendo agli ospitanti risparmi in risorse proprie. In Italia, invece, vi sono forti interessi a tenere in piedi le missioni internazionali, perché collegate alle attività delle aziende produttrici di armi e ai vertici militari collusi con le stesse nel favorirne gli affari a scapito della finanza pubblica. Le missioni militari sono quelle che giustificano il continuo, dissennato utilizzo dei nostri poligoni militari e la spendita di una montagna di soldi che circolano intorno al sistema poligoni. Le aziende che costruiscono armi e mezzi militari, i vertici delle Forze armate e il Ministero della difesa costituiscono un triangolo di interessi che si sorregge con i nostri soldi pubblici. Il tutto va, ovviamente, a scapito del sistema produttivo nazionale, entrato in crisi soprattutto per il moltiplicarsi di investimenti improduttivi, come possono essere considerati tutti quelli che riguardano la produzione di armamenti e di mezzi militari. Nell'insieme, il decreto-legge comprende oltre trenta diversi interventi militari all'estero, in più di venti Paesi diversi, senza contare le iniziative che si caratterizzano per l'impiego primario di strumenti non militari. A fronte di una simile complessità, sfuggono le ragioni di una diretta conversione in legge che, tra le tante cose, ha il sicuro effetto di sminuire il decreto-legge continui a disporre la proroga d'interventi militari che, quando non sono dannosi, sono quanto meno anacronistici. Malgrado ciò, il nostro Paese sembra aver bisogno di nuovi strumenti per fronteggiare altre emergenze, tanto da aver da ultimo disposto Triton, ancora un'altra operazione di monitoraggio del traffico marittimo. Superata dalle circostanze è la missione EUFOR Althea. La situazione della Bosnia-Erzegovina sembra già essere mutata, tanto da aver già sottoscritto nel 2007 l'accordo di stabilizzazione e associazione all'Unione europea. Stesso discorso vale per la proroga della missione Temporary International Presence in Hebron, che tutto sembra tranne che temporanea, risalendo a vent'anni fa. Veniamo alla partecipazione italiana alle operazioni militari di maggior scopo e portata, come l'International Security Assistance Force della NATO in

un finto ritiro per proseguire l'insensata presenza in una guerra, che è costata già 54 morti italiani e centinaia di vittime civili. Inoltre, non possiamo non chiederci quanti degli obiettivi posti alla base della United Nation Interim Force in Lebanon siano stati conseguiti, in modo da poter almeno intravedere Come poi non possiamo chiederci in che modo si sia giunti all'invio di ancora altri nostri uomini in Kurdistan e quale siano la natura, gli scopi e la durata di questo particolare impegno. Nelle presenti e prevedibili circostanze, è evidente come la partecipazione militare italiana alle missioni internazionali in generale, e in Libano e in Afghanistan in particolare, risponda al desiderio di ritagliare, attraverso l'impiego del nostro dispositivo militare, un ruolo internazionale confacente agli interessi delle *lobby* del traffico d'armi, legale e non, più che alle esigenze della popolazione italiana, costretta a veder bruciate tantissime risorse economiche a vantaggio di un immane sperpero di soldi pubblici per andare a sparare in giro per il mondo. E questo non deve farci dimenticare che spesso, oltre che uno spreco di denaro e di vite umane, le missioni internazionali in cui è coinvolta l'Italia contribuiscono addirittura a peggiorare la situazione, come è accaduto nei casi delle guerre in Iraq ed in Libia.

prima di entrare nel vivo del mio intervento e alla luce degli ultimi avvenimenti verificatisi a Milano, dove si è compiuta una vera propria strage, vorrei porgere il mio sostegno e la mia ammirazione a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine e ai militari che quotidianamente rischiano la propria vita, sacrificando la loro esistenza, per garantire a tutti noi la sicurezza di poter girare nelle strade del nostro Paese e sentirci sicuri e protetti. L'Italia non corre alcun rischio, il nostro Paese è sicuro: sono frasi degli ultimi mesi pronunciate dal ministro Alfano. Direi che possiamo stare veramente tranquilli se la nostra incolumità è affidata a questo Ministro. Orlando e Alfano si sono chiesti, alla luce della sparatoria nel tribunale di Milano, in che stato sia effettivamente il sistema di protezione e di controllo in Italia. Se un privato cittadino è riuscito a compiere una strage, mi domando un terrorista, una persona addestrata militarmente cosa mai avrebbe potuto fare. E stiamo parlando di un tribunale in una città come Milano. Vorrei, da cittadino e da parlamentare, che i ministri Alfano e Orlando venissero a riferire in Aula, o per lo meno facessero *mea culpa* davanti agli italiani. Forza Italia è una forza responsabile, che ha come unico obiettivo portare avanti riforme e provvedimenti che vadano a favore degli italiani. quindi, sottolineare, nel corso del mio intervento, alcuni aspetti critici del decreto-legge. Dobbiamo innanzi tutto rimarcare, con forza e nitidezza, che il terrorismo è una piaga urgente e reale, che non permette perdite di tempo e azioni deboli, poco chiare, ma necessita di reazioni ferme e decise. Si parla della vita di milioni di persone, dei nostri cari. Signor Sottosegretario, Sottosegretario, la ringrazierei se mi desse la possibilità di continuare a svolgere il mio intervento e bloccasse, invece, la sua chiacchierata con la collega nel banco sottostante Ma capisco che non è interessato a tale argomento. La prego, signor Presidente, di richiamare il Sottosegretario Cassano all'ascolto. Dobbiamo, innanzitutto, rimarcare con forza e con nitidezza che il terrorismo è una piaga urgente e reale, che non permette perdite di tempo e azioni deboli, poco chiare, ma necessita di reazioni ferme e decisive. Si parla della vita di milioni di persone, dei nostri cari, delle nostre famiglie e dei nostri figli. Quando si parla dei nostri figli, automaticamente il pensiero va a quello che sarà il nostro futuro: giovani di altri Paesi, solo apparentemente lontani da noi, sono pronti a sacrificare la loro vita,

L'Occidente sino ad oggi ha solo dimostrato di non avere compreso fino in fondo quelle culture, quelle radici, quelle convinzioni che appartengono ad ognuno di quei popoli.

Questo decreto-legge si compone di due parti. La prima riguarda le misure antiterrorismo e la seconda tratta della proroga delle missioni di pace internazionale cui partecipa l'Italia. Quanto alla lotta al terrorismo, le misure adottate sembrano andare nella giusta direzione, perché mirano a potenziare i servizi di *intelligence* e a rafforzare il controllo del territorio nazionale. Mi riferisco - ad esempio - alle disposizioni che introducono nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, in particolare alle norme che prevedono la reclusione per chiunque si arruola in gruppi terroristici e per chi organizza i viaggi deputati a tale scopo. Inoltre, dal momento che nel mondo contemporaneo la propaganda terroristica avviene anche e soprattutto mediante la comunicazione via *web*, è previsto che vengano costantemente monitorati tutti i siti utilizzati per finalità terroristiche, con l'eventualità che i contenuti ritenuti illeciti vengano rimossi dal sito. Infine, non è di poco conto che il procuratore nazionale antimafia assuma anche le funzioni di procuratore nazionale antiterrorismo. In realtà, le misure contenute nel decreto-legge, seppure importanti ed utili, non bastano. Non bastano perché il terrorismo non attiene unicamente alla sfera nazionale, ma è un problema di carattere transnazionale. Per queste ragioni, l'Europa ha un ruolo cruciale e decisivo che, tuttavia, sembra si rifiuti di svolgere. L'Unione europea dovrebbe adottare delle misure urgenti in considerazione dell'estremo pericolo che minaccia l'intero continente. In più, dovrebbe tutelare con misure straordinarie la nostra penisola, proprio perché geograficamente più vicina alle frontiere del Nord Africa.

Sappiamo, infatti, che attualmente il bacino del Mediterraneo è teatro di conflitti e di attività terroristiche. I Paesi dell'Africa del Nord stanno attraversando un momento molto delicato: l'instabilità politica e il collasso delle istituzioni sono fattori che favoriscono l'avanzata di gruppi terroristici all'interno dei propri territori e costituiscono una vera e propria minaccia alla sicurezza internazionale. Si tratta di una situazione che mette a rischio i principi stessi di libertà e democrazia su cui si basa l'Unione europea. Di ciò le istituzioni europee dovrebbero farsi carico, con l'elaborazione di una strategia di politica estera che dia una risposta adeguata all'attuale situazione del Mediterraneo e del Medio Oriente, avendo riguardo in particolare all'Italia. Quindi, l'Europa deve essere decisa e chiara nelle sue scelte e nelle azioni da intraprendere. Accanto a noi - e lo dico da italiano e da siciliano - sono in atto delle vere e proprie guerre e l'Italia da sola non può farcela. Immagino un'Europa che non ci imponga solo restrizioni economiche, ma che ci faccia sentire parte di un progetto più ampio e non ci lasci soli. Faccio un piccolo passo indietro e ritorno alle mie parole sul tentativo ostinato di non voler capire che i popoli dei Paesi arabi hanno una propria identità in quanto sono e si sentono Nazione.

imponendo regole e privando loro di una propria identità di popolo e Nazione, impedendo il concetto di autodeterminazione che è proprio di ogni popolo. La seconda parte del decreto-legge dispone la proroga delle missioni di pace all'estero. Sono favorevole, perché con queste misure manteniamo il nostro impegno e il nostro contributo alle attività di sostegno alla pace portate avanti dalle organizzazioni internazionali. Per questo dovremmo sgombrare il campo da ogni polemica interna, che avrebbe l'unico risultato di indebolire l'immagine e la credibilità dell'Italia nei confronti del mondo. Non serve, almeno su questo punto, dividerci: cerchiamo di agire insieme per rendere effettivo quel principio di libertà che tutti indistintamente, almeno a parole, sbandieriamo a gran voce. Lo dobbiamo ai nostri militari, che devono avere alle spalle un Paese unito, e che stia dalla loro parte, e uno Stato che tuteli le regole di ingaggio e rispetti i principi della Costituzione. Al riguardo, condivido la *ratio* dell'articolo 13, che subordina la prosecuzione della missione antipirateria Atalanta agli sviluppi della vicenda dei due marò. Vorrei sviluppare un'ultima riflessione,

dandovi qualche specifica e qualche numero. Per esempio, in Europa l'Italia partecipa a diverse missioni: una nei Balcani,

opera su tutto il Medio Oriente per 519.000 euro. Scendendo, ci sono altre missioni per circa 2 milioni di euro e arriviamo in Africa.

Considerate che, solo per la voce «Contratti di assicurazione, trasporto e realizzazione infrastrutture» paghiamo 73.457.600 euro. Signori: realizzazione di infrastrutture! Signor Presidente, ma dove? ma dove? Cominciamo qui a parlare di attualità: se discutiamo di infrastrutture, perché in questo momento dobbiamo parlare di infrastrutture che vogliamo

vero: il terrorismo delle aziende e di chi ha amministrato, di chi ha costruito quei ponti che stanno venendo giù come ruscelli di sabbia! Bisognerebbe parlare di questo. Bisognerebbe parlare della ristrutturazione delle scuole che stanno cadendo. Poco fa c'era il Ministro, ma intanto non

L'uomo oscuro che fa il Presidente del Consiglio, che viene a raccontarci che c'è un tesoretto in Italia e non sa come spenderlo, oggi spende un miliardo di euro per mandare i nostri soldati in giro per il mondo a portare guerra.

Allora o lei si dimette o trova una soluzione immediatamente, perché i cittadini di quel territorio, che hanno subito danni oggettivi per la maledetta guerra in Libia, non sono stati risarciti di nulla.

antiterrorismo parliamo? Fino ad ora è andata benissimo, ma non è detto che continui così. Arrivano le persone, vengono prese dal porto e portate in quei centri

Siete convinti che l'immigrazione non sia correlata a tutto quello che avviene nel mondo e alle guerre. Siete convinti sia il frutto della casualità, mentre è frutto delle bombe che anche voi, italiani, andate a far esplodere nelle Nazioni del mondo. Davanti a questo scempio, signor Presidente, diremo con fermezza un no deciso e concreto. Abbiamo anche questa volta presentato emendamenti e vedremo se avrete la dignità

Un vergognoso sistema affaristico è emerso per le grandi opere, sollevando la solita ipocrita reazione di un Governo che, proprio in quel sistema, affonda le radici principali del suo consenso. La musica non cambia per le opere pubbliche ordinarie, per cui l'attuale sistema di potere, monopolizzato dai soliti partiti dei "giovani vecchi renziani", ormai sparsi in ogni dove tra destra e sinistra, nonostante i trionfali annunci propagandistici, non è in grado di assicurare le condizioni minime di sicurezza nemmeno ai bambini delle scuole. È una vergogna, il fallimento totale di una classe politica e di un sistema di amministrazione della cosa pubblica e dei lavori pubblici che deve essere radicalmente cambiato. L'invito è quello - per una volta - di pensare al futuro dei nostri ragazzi e non alle casse di qualche imprenditore compiacente o ai voti per le prossime elezioni. I cittadini ormai hanno compreso che non possono avere alcuna fiducia nei partiti della vecchia politica, gestiti oggi da giovani dall'animo ancor più vecchio di quelli che li hanno preceduti.

raggiunta con 165 treni merci al giorno. Dai dati ufficiali Eurostat, il numero di convogli nel 2010 è stato invece di 65, per cui siamo lontanissimi dalla saturazione.

Da ulteriori riflessioni poi, basate sempre su dati reali assunti dalle banche dati, si giunge all'amara considerazione che le Ferrovie hanno la consuetudine a sovrastimare queste progettualità e sempre con un fattore di circa 15 volte maggiore. Ancora una volta, supportato dai dati, posso affermare che quella del terzo valico è un'opera inutile, dove i costi superano di gran lunga gli inesistenti benefici. Si producono analisi oniriche, fantastiche, per giustificare quanto di più irrazionale si è progettato ed ora si vuole realizzare. I cittadini ne sono coscienti, l'inganno è svelato. Ognuno di noi, con la diligenza del buon padre di famiglia - quella che manca a questo Governo - sa che il Terzo valico dei Giovi è costruito ad unico beneficio di *lobby* che vogliono arricchirsi. Per questo motivo - e chiudo - domani sarò ad Arquata Scrivia per vigilare sull'ennesimo tentativo di effettuare espropri. L'ultima volta hanno cercato di manganellarmi; stavolta, magari, fatemi una fotografia, così ci riuscite.

che, all'articolo 7, parla di detrazioni che vanno dai 900 ai 450 euro per gli abitanti in affitto in alloggi di edilizia sociale.

Signor Presidente, colleghi, tra qualche settimana commemoreremo il ventesimo anniversario del genocidio di Srebrenica: una tragedia che - lo ripetiamo ogni anno - dovrebbe essere un monito per qualcosa che non si deve più ripetere. Eppure, proprio pochi giorni fa, l'UNICEF ha parlato di una nuova Srebrenica, in riferimento alla sanguinosa offensiva dell'ISIS nel campo profughi di Yarmouk, alle porte di Damasco. Dinanzi a questa vergogna mi chiedo cosa stiamo facendo. Sono certamente da apprezzare l'intervento del ministro Gentiloni sul tema e lo stanziamento dei fondi per un corridoio umanitario. Ma l'Italia deve farsi sentire con forza nei contesti internazionali, per sollecitare un'azione incisiva che vada al di là dello sgomento generale. Oggi a Yarmouk 3.500 bambini vivono intrappolati senza cibo né acqua e la popolazione è soggetta ad una brutale violenza assassina. Non possiamo permetterci una memoria così breve da rimanere inerti a guardare quest'ennesima tragedia umanitaria. Sollecito, dunque, il Governo del mio Paese a prendere adeguate iniziative. **Per Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un evento accaduto in Sicilia il 10 aprile, che ha avuto risonanza nazionale. Si tratta dell'ennesimo cedimento strutturale di un viadotto dell'autostrada, questa volta causato da una frana collinare, sulla A19 Palermo-Catania, al km 57,500 del viadotto Himera. A seguito di tale cedimento, la Sicilia è letteralmente paralizzata e divisa in due, anche in considerazione del fatto che alcune zone interne sono già da tempo isolate, nella zona delle Madonie, per le frane provocate dal maltempo delle ultime settimane. In queste ore - al di là delle opportune e inderogabili verifiche che dovranno essere fatte per stabilire gli eventuali livelli di responsabilità ed omissioni a cui ricondurre l'evento - sono state effettuate le prime rilevazioni tecniche e, secondo quanto è dato apprendere, è emerso che il viadotto Himera è destinato a crollare per cedimento naturale o perché verrà abbattuto e poi ricostruito a causa del danno irreparabile. Ancora ieri, un incontro congiunto qui a Roma tra ANAS, Regione, assessorati regionali coinvolti, tecnici e Dipartimento della protezione civile ha avuto lo scopo di definire il calendario che porterà al ripristino dei collegamenti fra Palermo e Catania e di fare una prima stima e di fare una prima stima dei costi per il ripristino del tratto autostradale. Secondo quanto è emerso, un percorso alternativo dovrà essere individuato entro un paio di mesi, con un ulteriore aggravio di costi e tempi per i cittadini fino a tale data. È chiaro che ciò che è accaduto è l'ulteriore conferma di quanto sia fondamentale fare una mappatura su tutto il territorio della condizione della viabilità stradale e ferroviaria e, se questo vale per tutto il nostro Paese, tanto più per la Regione Siciliana, che rischia un ulteriore isolamento grazie oltre alle ovvie determinazioni da assumere per fare piena luce su questo ennesimo episodio ed accertare le eventuali omissioni e responsabilità sul piano amministrativo, tecnico e disciplinare quali provvedimenti intenda adottare, di concerto con i soggetti interessati, per prevenire il verificarsi in futuro di simili inaccettabili situazioni, che mettono a rischio la vita dei cittadini. se non ritenga inoltre opportuno, per quanto di competenza, sollecitare i soggetti interessati per prevedere il potenziamento della viabilità su ferro e l'implementazione della rete infrastrutturale secondaria della Regione e soprattutto se non ritenga opportuna